Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 29 giugno alle ore 14 per la votazione relativa all'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

sulla partecipazione di Taiwan a organizzazioni internazionali. Ha facoltà di parlare il senatore Malan per illustrarla. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, Taiwan è la ventiduesima economia del mondo, è il diciottesimo *partner* dell'Unione europea per interscambio,

che lavorano in particolare per la sicurezza e la salute internazionale e, dunque, nell'interesse della collettività, della comunità internazionale e della popolazione taiwanese.

a considerare attivamente, insieme ai *partner* dell'Unione europea, compatibilmente con gli accordi internazionali già sottoscritti, le modalità per consentire la partecipazione come osservatore di Taiwan ai contesti internazionali che ho citato, ai quali va aggiunta l'Assemblea mondiale della sanità, al fine di migliorare la sicurezza collettiva, i rapporti internazionali

una isola dalle travagliate relazioni internazionali, soprattutto con la stessa Cina continentale.

tra le 22 economie più importanti del mondo; è il diciottesimo *partner* dell'Unione europea per volumi di interscambio e con l'Italia intrattiene relazioni culturali, commerciali e industriali piuttosto interessanti.

nel breve giro di pochi mesi, Taiwan ha dovuto subire, verosimilmente a causa di irresistibili pressioni da parte di Pechino, il mancato invito a prendere parte ad alcune attività a cui era già stato invitato

della sanità è stata pretesa e ottenuta da parte del Governo cinese dopo otto anni di partecipazione, tra l'altro molto apprezzata sia per l'apporto scientifico che per le efficaci cooperazioni.

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, la mozione presentata a dicembre 2016 è stata riformulata, con un testo 2, ancorché ulteriormente riformulato in un testo 3, escludendo intere parti nelle premesse e riformulando il dispositivo. È assai probabile che ci sia stato qualche ispiratore che ha consigliato il Governo e, a cascata, il senatore Sangalli, e questo ce ne dispiace. Occorre riconoscere, ad esempio, che nel 2013 Taiwan era stata invitata a partecipare alla 38a assemblea dell'ICAO e che si attendeva che tale invito fosse rinnovato anche all'ultima assemblea, la 39a, svoltasi a Montreal lo scorso settembre, proprio a motivo del positivo precedente del 2013 e del fatto che le materie e le competenze proprie dell'ICAO sono di carattere tecnico e riguardano direttamente il destino di centinaia di milioni di passeggeri. Invece, diversamente dalle attese, lo scorso anno Taiwan non è stata invitata alla 39a assemblea. Evidentemente motivazioni di natura completamente estranea alle finalità e ai doveri dell'ICAO hanno condizionato, in modo tanto invasivo, le sue funzioni e responsabilità così strettamente connesse alla vita e alla sicurezza di tutti coloro che utilizzano il trasporto aereo. Eppure non è irrilevante sottolineare che dagli scali aerei e portuali dell'Isola transitano, annualmente, 60 milioni di persone. Ci spiace che la Cina prosegua con questo ostracismo nei confronti della democratica Taiwan e dei suoi 23,5 milioni di abitanti in nome del mantra "One China policy". Un ostracismo che è stato confermato anche nelle recenti settimane con la gravissima esclusione di Taiwan dall'Assemblea mondiale della sanità che si è tenuta a Ginevra nell'ultima decade del mese di maggio. La Cina ha preteso e imposto l'esclusione di Taiwan da tale Assemblea per proprie ragioni politiche, pubblicamente dichiarate, di avversione al Governo taiwanese democraticamente eletto nel 2016. Una democrazia - lo sottolineo - tra le più progredite dal punto di vista dei diritti civili, politici, religiosi e sindacali. E la motivazione politica dell'ostracismo contro Taiwan è talmente evidente - e perciò inaccettabile - per il fatto che negli ultimi otto anni, dal 2009 al 2016, Taiwan ha sempre partecipato da osservatore a questo organo decisionale dell'OMS dando un valido e apprezzato contributo sanitario e scientifico, visto che virus, malattie ed epidemie non si fermano innanzi ai confini nazionali né a regimi di qualunque colore politico. È gravissimo questo ostracismo politico, ma ancor più grave che l'Assemblea mondiale della sanità e l'Organizzazione mondiale della sanità (che quest'anno hanno fatto forse più notizia per le scandalose spese per viaggi e soggiorni di propri funzionari, direttore generale incluso) si siano prestate a questi giochi, visto che dovrebbero essere apolitiche e che nel loro atto costitutivo stabiliscono di operare - oggi dobbiamo dire «dovrebbero» - per gli esclusivi obiettivi della tutela e della promozione della salute del genere umano, anche attraverso la sicurezza alimentare, per perseguire il benessere dell'umanità, al di fuori e al di sopra di ogni motivazione razziale, religiosa, politica ed economica. Solo la caparbietà e la responsabilità del Governo di Taipei ha fatto sì che a Ginevra si recasse ugualmente il Ministro della sanità che ha avuto, fuori dalla sede dell'Assemblea, incontri bilaterali con i colleghi di trentuno e con i vertici di ventotto organizzazioni internazionali che operano nel campo della salute e della cooperazione. Per i predetti motivi, come parlamentari della Lega Nord che hanno sottoscritto la mozione, chiediamo al Governo di coordinarsi con gli altri Esecutivi dell'Unione europea e di adoperarsi affinché Taiwan - lo sottolineo, ventiduesima economia al mondo

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, credo non sfugga a nessuno l'elemento di delicatezza dei rapporti tra Taiwan e la Repubblica Popolare Cinese, quindi è all'interno di tale delicato equilibrio che va a inserirsi quale abbiamo apprezzato la riformulazione proposta dai proponenti d'intesa con il Governo. È necessario un approccio di tipo pragmatico, cercando di fare lavorare la diplomazia che spesso ha tempi lunghi, ma consente di mantenere quel delicato equilibrio che credo sia necessario nei rapporti tra Taiwan e la Repubblica Popolare Cinese. In questa prospettiva, esprimiamo come Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico progressista il nostro voto favorevole

anche se - questo è il mio punto di vista - ancora non ci riteniamo completamente soddisfatti, perché siamo fondamentalmente convinti che nei confronti di questo importante Paese, tra l'altro *partner* ci siano ancora notevoli pregiudizi e ostracismi. Ci rendiamo conto dei condizionamenti che vengono dalle politiche internazionali e anche dai rapporti che giustamente il nostro Paese e l'Unione europea hanno con la Cina continentale, Grazie

e democrazia e di voler intrattenere, in particolare con l'Italia, una corsia preferenziale dal punto di vista dei rapporti economici e dei rapporti bilaterali.

il presidente Trump ha successivamente smentito le sue dichiarazioni, costringendo probabilmente il senatore Malan a riformulare questa mozione, che oggi ha cambiato completamente significato. Questa richiesta al Governo per noi non vuol dire assolutamente nulla, né tanto meno riteniamo che possa sostenere in qualche modo il nostro interesse nazionale, dato che l'interscambio commerciale con Taiwan di certo non risentirà dell'approvazione di questa mozione. Allo stesso tempo, non riteniamo che il Parlamento debba esprimersi su un tema che riguarda la politica estera di Taiwan e la sua eventuale partecipazione agli organismi internazionali indicati. Per questo motivo, il Movimento 5 Stelle si asterrà e si augura che in futuro si eviti di discutere di mozioni a nostro avviso inutili come questa. che si parlasse un po' di più del CETA, che oggi verrà esaminato in Commissione affari esteri e che passerà successivamente all'esame dell'Aula, di cui nessun giornale sta parlando; i cittadini sono ignari di quello che questo trattato con il Canada comporta. Ricordo inoltre che da mesi il Movimento 5 Stelle attende la calendarizzazione di una mozione sulla politica estera del nostro Paese, che riguarda Afghanistan, Siria e Libia e che a nostro avviso è sicuramente più importante per gli italiani della partecipazione di Taiwan agli organismi internazionali. Ribadisco quindi che il Movimento 5 Stelle si asterrà.

con il testo 1 e che rimane del tutto immutata nel testo 2 è quella di chiedere al Governo un impegno a consentire la partecipazione di Taiwan ad alcuni contesti multilaterali, di cui ho già parlato nel mio primo intervento. Mi riferisco a quello sull'aviazione civile, all'organismo delle Nazioni Unite che si occupa di clima, all'Interpol e ad altri organismi ad altri organismi internazionali, dove è senza dubbio interesse della comunità internazionale e della popolazione taiwanese continuare ad avere questa collaborazione. mozione che sono state cambiate, non si sono sottolineati alcuni punti di questa vicenda che riguarda Taiwan, allo scopo evidente di raggiungere un accordo tale che permettesse di approvare la sua approvazione, avremo un impegno da parte del Governo a favorire la partecipazione di Taiwan a questi organismi internazionali. Non è certo oggi che viene approvata, ratificata o incoraggiata la *One China policy*, frutto di decenni di lavorio, di contatti e di pressioni da parte delle parti in causa. Il tutto ha avuto origine quando la Repubblica popolare cinese, che era stata esclusa dalle Nazioni Unite fino agli anni '70, venne inclusa per iniziativa della presidenza Nixon degli Stati Uniti. Questa era la cosa giusta da fare, perché lasciare lo Stato più popoloso del mondo al di fuori delle Nazioni Unite sarebbe stato davvero un controsenso. Certo, si prese una decisione assai discutibile, ed è questa la motivazione per cui ho sempre fatto parte del gruppo di amicizia parlamentare fra Italia e Taiwan: quella di mettere al contempo fuori dalle Nazioni Unite (e non solo di darle un riconoscimento inferiore) la Repubblica di Cina, il cui territorio coincide di fatto con l'isola di Taiwan, più alcune piccole isole ad essa vicine; un Governo che era in continuità con la potenza della

più di qualsiasi altro Paese, persino più dell'Unione sovietica. È stato, altresì, il Paese che più a lungo ha combattuto contro le potenze dell'asse iniziando il suo il suo confronto con il Giappone, a causa dell'invasione giapponese, molto prima dell'inizio della Seconda guerra mondiale. Metterlo completamente fuori, senza tutela alcuna, Grazie

di dare a questo Paese almeno l'appoggio per partecipare a quegli organismi internazionali che servono non al prestigio taiwanese, ma alla sicurezza internazionale, alla tutela delle persone che da tutto il mondo, inclusa la

nella classificazione economica internazionale ci si ricorda di molti aspetti di questo Paese. Faccio riferimento a due marchi industriali: Acer e Asus. Sono i più grandi produttori di componentistica per informatica del siamo di fronte a un Paese di altissimo *standard* tecnologico che, nel giro di pochi decenni, è passato dell'essere un Paese povero e agricolo a essere prima un Paese industriale e e manifatturiero e poi un Paese ad altissima produzione tecnologica. Oggi oltre il 65 per cento della popolazione di Taiwan, che ha un reddito medio molto elevato, è occupata nei servizi ad alto valore aggiunto. Stiamo parlando di un Paese economicamente importante, anche se certamente non importante per noi quanto la Repubblica popolare cinese, perché è un Paese le cui dimensioni, il cui ruolo internazionale e nella

Grazie ricordato che Formosa, diventata poi Taiwan, era la rappresentante nelle Nazioni Unite dell'intera Cina e non era rappresentata la Cinapopolare. È stata una storia che si è evoluta molto.

nel 1992 con l'accordo cosiddetto 1992 Consensus si realizza quello che viene chiamato il One China Policy: il riconoscimento di un'unica Cina non come Paese o come Nazione, ma come dati culturali e storici. Sulla base di questo accordo, l'allora presidente taiwanese sviluppò un intenso rapporto con la Repubblica popolare cinese. Pertanto, da Paese minacciato di un'invasione prossima della Cina, si passa ad un Paese che, pur non avendo relazioni diplomatiche se non con Paesi non non significativi nello scacchiere internazionale, a parte Città del Vaticano, intrattiene rapporti tenuti essenzialmente tra rappresentanze commerciali che assumono il valore di rappresentanze diplomatiche.

amministrative, del Parlamento e il cui Presidente è eletto dal popolo. Siamo in una situazione che nell'ambito dei rapporti multilaterali va guardata con molta attenzione. Mi dispiace per chi la sottovaluta, ma la posizione di questo Paese è strategica non soltanto nel rapporto con la Cina. Teniamo conto che i rapporti con la Cina sono tesi dal punto di vista formale, ma dal punto di vista sostanziale sono molto proattivi; ci sono oltre mezzo milione di cinesi

La politica estera è fatta di segnali, di accordi, di trattati, di costruzione di un consesso, sapendo strategicamente quali possono essere le minacce nel medio e lungo termine. Mi dispiace che quando si esce dal confine del proprio paesello tutto il mondo diventa misterioso, ma qualche volta serve anche documentarsi su questa parte del mondo e sui potenziali rischi che in mancanza di un processo di distensione e di accordo potrebbero esserci. Voteremo pertanto a favore della mozione che unitariamente abbiamo partecipato a scrivere;

come ha prodotto effetti commerciali rilevanti fra i due Paesi, possa determinare effetti politici rilevanti nell'entrata di Taiwan a pieno titolo nei diversi consessi ed organismi internazionali in cui ha titolo ad essere rappresentata non contro la Cina, ma nell'ambito di quella cultura di avvicinamento tra la Repubblica popolare cinese e Taiwan. Per tale motivo, il voto del Gruppo del Partito Democratico

Signor Presidente, colleghi, il presente intervento si colloca sulla scia di altri già da me effettuati, così come da tanti altri colleghi. Invero, sotto i riflettori, di volta in volta, sono state le politiche industriali di grandi gruppi e le prospettive occupazionali dei lavoratori dei siti interessati da operazioni di esternalizzazione e dunque numerosi atti di sindacato ispettivo, e non, sono stati presentati al fine di conoscere la fattibilità e la concretezza delle operazioni stabilite dalle varie aziende coinvolte. Oggi porto all'attenzione le intenzioni del colosso delle telecomunicazioni Wind Tre così come accennate dai sindacati durante il tavolo indetto per la presentazione del piano industriale della nuova compagnia sorta a seguito delle note operazioni di fusione Wind Tre. In ballo il *customer care* ex H3G operativo nelle sedi di Palermo, Roma, Cagliari e Genova. Pertanto, *in primis* le forti preoccupazioni per il futuro dei lavoratori coinvolti riguardano proprio la salvaguardia dei posti di lavoro. Dalla stampa si apprende come non siano ancora pervenute le risposte attese già da diversi mesi, tanto da portare le segreterie nazionali di vari sindacati come FISTel-CISL, SLC-CGIL e Uilcom-UIL, con un comunicato nazionale del 22 maggio ultimo scorso, a ribadire la necessità di avere maggiore chiarezza sulla tenuta del perimetro aziendale complessivo,

che la fusione venga scaricata interamente sui lavoratori, sono state portate alla luce anche dalla segreteria nazionale UGL Telecomunicazioni. originano dalla decisione di Wind Tre SpA di procedere all'esternalizzazione del servizio di *customer* *care* ovvero il servizio svolto dal *contact center* ex H3G, dove i lavoratori impiegati ammontano a circa 910, divisi nelle quattro sedi di Palermo, Roma, Cagliari e Genova. Del resto, non sono pervenute informazioni, neppure marginali ed ufficiose, circa il nome dell'azienda a cui sarà affidato il servizio in *outsourcing.* Al riguardo, pertanto, nutro le stesse perplessità delle suddette organizzazioni sindacali; l'esperienza maturata in casi analoghi o comunque similari ha mostrato come operazioni del genere si siano rivelate fallimentari. Ovviamente nel breve periodo non vi è alcun rischio, dato che in caso di cessione di ramo d'azienda i dipendenti traghettano, con il loro contratto di lavoro, all'azienda che acquisisce. Tuttavia, non dimentichiamo quanto accaduto l'anno scorso con il gruppo Almaviva, così come in altri casi di esternalizzazione. Concludo ricordando che giovedì prossimo, il 29 giugno, è previsto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche sociali, un tavolo politico con la speranza che in tale incontro venga presentato un piano industriale che investa davvero sul capitale umano non una mera operazione finanziaria. Quindi, ovviamente, mi auguro che ci sia la possibilità di salvare i posti di lavoro in bilico.

in provincia di Treviso. Lì si lavora ancora con le catene di montaggio a tapparella, con il ritmo vincolato. Da anni i delegati sindacali contestano ritmi di lavoro troppo intensi. Non è una fantasia: in quell'impianto sono stati riconosciuti dall'INAIL oltre 181 casi di malattia professionale legata ai movimenti ripetitivi su 700 unità lavorative. Quindi, parliamo di livelli di morbilità incredibili. Il delegato FIOM della Electrolux, Augustin Bruno Breda, è diventato un esperto dei calcoli legati ai tempi di lavorazione.

da un *detective* e scopre che, invece di passare tutto il tempo accanto all'ammalato, Bruno va anche a fare la spesa a va alla posta a ritirare la pensione. Per questo gli contesta un cattivo uso della legge n. 104 e lo licenzia.

hanno fatto ventisette ore di sciopero. E chi sa quanto guadagna un operaio metalmeccanico si rende conto di cosa significhino ventisette ore di sciopero per questi lavoratori, che scioperano per difendere colui che li rappresentava colui che li rappresentava e che è stato licenziato. Io sto presentando un'interrogazione, nella quale chiedo al Ministro del lavoro e al Ministro della salute cosa intendano fare: per questa situazione specifica di Breda, ma anche per il livello di malattie professionali in quell'impianto: 181 persone su 700 sono un livello di incidenza inaccettabile in una società che una volta si definiva occidentale ed evoluta. Questo volevo rappresentarvi, affinché sappiate che in Italia abbiamo questo tipo di realtà, che è ancora assolutamente esistente ed è fatta di sofferenza reale e perché rispetto a questo noi assumiamo una posizione chiara per evitare che la gente fuori pensi che noi siamo assolutamente distaccati da queste realtà e da questo livello di vita reale.

Grazie